L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Presidente, il testo proposto dalla Commissione all'Assemblea prevede il distacco del Comune di Sappada dalla Provincia veneta di Belluno e la conseguente aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della Provincia di Udine. Il testo proposto, approvato dalla Commissione il 2 febbraio 2016, si inserisce nel procedimento di cui all'articolo 132, comma 2, della Costituzione, che prevede che Province e Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra quando la richiesta dell'ente interessato, previo *referendum* popolare e sentiti i consigli regionali, sia approvata con legge della Repubblica. Appare utile ricordare che la disposizione costituzionale non distingue in base alla natura ordinaria o speciale della Regione, tema che assume particolare interesse per il caso in esame, in quanto il Comune di Sappada chiede il distacco dalla Regione Veneto e l'annessione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui Statuto è stato approvato con legge costituzionale. La necessità di una legge costituzionale

laddove, definendo le caratteristiche dell'atto normativo con cui si dispone l'aggregazione del Comune ad altra Regione, si stabilisce che tale atto debba essere una legge ordinaria. Tale lettura è confermata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007 riguardante il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e l'aggregazione alla Valle D'Aosta. le disposizioni del citato articolo 132 si riferiscono a tutte le Regioni, senza deroghe alla procedura qualora una delle Regioni interessate sia dotata di uno statuto approvato con legge costituzionale. È opportuno ricordare che nel 2008 il Comune di Sappada ha svolto con esito ampiamente favorevole il prescritto *referendum* e che la richiesta soddisfa i requisiti, previsti dalla legge, di continuità geografica, omogeneità economica e sociale

Posso anche sbagliarmi, ma mi pare che nelle ultime due legislature siamo riusciti a rispondere solo ai cittadini dell'Alta Valmarecchia, spaccata in più zone, una in Provincia di Arezzo e l'altra sul versante emiliano, e abbiamo ricomposto l'unità della valle. Dovremmo aver finito i percorsi di Cinto Caomaggiore, Magasa e Valvestino, però mancano ancora i provvedimenti governativi, cioè l'atto cui deve provvedere il Governo e noi speriamo che anche Sappada possa vedere la fine la fine di questo percorso. Vorrei ricordare che i provvedimenti di competenza locale, già esauriti, si sono definiti per l'altopiano di Asiago e i sette Comuni; Pedemonte e Casotto, Comuni che da sempre hanno gravitato nell'area trentina, appartenuti fino al 1918 al Tirolo storico e fino al 1929 alla Provincia di Trento,

torrente Cismon, per cui nell'area trentina. Addirittura per passare da una valle trentina a un'altra valle trentina, cioè dalla Valsugana al Primiero, si attraversa questa piccola gola che però si trova nelle

che la nostra Costituzione ha individuato e ha posto come base la libertà dei cittadini di riconoscersi nell'ente che più ritengono opportuno. Questa libertà spesso non è rispettata dagli stessi enti, che scavalcano addirittura la Costituzione, perché la nostra Carta fondamentale stabilisce che la maggioranza degli abitanti di un Comune

reca la proposta di istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta - per la durata di dodici mesi - sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto, centro di accoglienza per minori disagiati sottoposti alla vigilanza del tribunale, con annessa cooperativa agricola. Prima di procedere all'esame del provvedimento è opportuno dare conto, seppure sinteticamente, dei fatti sottesi alla proposta di inchiesta, rinviando per ogni approfondimento alla dettagliata relazione del La cooperativa agricola Il Forteto, comunità di recupero per minori disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni Settanta, culminata nel 1985 con una prima condanna definitiva dei cofondatori e conclusasi nel 2016 con un'ulteriore condanna (non ancora definitiva, ma confermata in sede di appello) a circa sedici anni di reclusione per gli stessi fondatori. Nonostante i gravissimi capi di imputazione, nel 1997 uno dei cofondatori risultava ancora a capo della comunità

l'Italia è stata condanna nel luglio 2000 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - adita dalle madri alle quali i minori erano stati tolti - a pagare una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali. È necessario segnalare all'Assemblea che la situazione della cooperativa è stata già oggetto di attenzione da parte delle istituzioni: da un lato, da parte della Regione Toscana, attraverso l'istituzione di ben due Commissioni di inchiesta (che hanno depositato le proprie relazioni finali nel 2013 e nel 2016) e, dall'altro, da parte del Ministero dello sviluppo economico

Passando al merito del disegno di legge, il testo consta di nove articoli. L'articolo 1 prevede che sia istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui predetti sui predetti fatti accaduti presso la comunità Il Forteto. I compiti della Commissione, enunciati nello stesso articolo 1, sono poi puntualmente indicati nell'articolo 2. La Commissione è chiamata ad accertare i fatti e le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità Il Forteto, anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità; nonché a verificare i presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura Il Forteto inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento. Il disegno di legge attribuisce poi alla Commissione il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

ho cercato veramente di capire e di far capire agli altri che in quella cooperativa qualcosa non aveva funzionato e che, nonostante il fondatore

ha sempre saputo e detto in qualche modo che le cose non andavano. Comprendo che la cooperativa agricola

È vero che è stato anche un luogo in cui diversi personaggi andavano a fare campagna elettorale,

Grazie,

appoggiato la richiesta di urgenza. È stato un percorso lungo, io vi ho stressato al massimo delle mie capacità per portare il provvedimento

Grazie, credo che la vicenda della comunità Il Forteto, sulla quale sinceramente non esistono aggettivi adeguati per descriverne l'enormità, debba essere

Roberto Fiesoli. Misura cautelare disposta dall'allora magistrato Carlo Casini. Nel giugno del 1979 Fiesoli torna in libertà. Il giorno stesso il tribunale dei minori assegna, incredibilmente, al Forteto un bambino affetto da sindrome di Down: una chiara sconfessione della misura cautelare disposta da Casini. Nel 1980 un consigliere regionale della Democrazia Cristiana presenta una interrogazione per chiedere informazioni sul Forteto, sollevando dubbi concreti sulle pratiche condotte nella comunità e ipotizzando alcune forme di plagio. Ma gli affidi da parte del tribunale dei minori di Firenze proseguono senza sosta. Nel 1985 viene emessa una sentenza di condanna per maltrattamenti e atti di libidine nei confronti di Fiesoli e del suo vice Goffredi. Nonostante la sentenza, il rapporto di collaborazione tra tribunale dei minori e comunità del Forteto non si interrompono mai. Andiamo al 1999. «Il Mulino» pubblica il primo libro sul Forteto e ne seguiranno molti altri. Nel 2000 la Corte europea dei diritti dell'uomo emette una sentenza di condanna a carica dello Stato dopo il ricorso di una madre che aveva visto affidare i propri figli Vi si legge: «Questa situazione e i precedenti penali di Fiesoli e Goffredi avrebbero dovuto indurre il tribunale dei minori ad esercitare una maggiore sorveglianza riguardo al controllo dei bambini all'interno del Forteto, che non sembra sottoposto a un effettivo controllo da parte delle autorità competenti». Ma gli affidi continuano e, anzi, nel corso degli anni successivi numerosi sono stati gli attestati di stima, i riconoscimenti istituzionali, le iniziative a sostegno del Forteto e - soprattutto fiumi di denaro di finanziamenti pubblici: dalle visite istituzionali e politiche di esponenti del centrosinistra a quelle di piacere (pranzi o spesa nella cooperativa) di alcuni magistrati, dalle presentazioni di libri di Fiesoli, alle ospitate pubbliche dello stesso Fiesoli (la più eclatante nel novembre 2011 a Palazzo Vecchio). E fino al 2009 il tribunale dei minori ha continuato implacabilmente ad inviare ragazzi disagiati al Forteto. Nel dicembre del 2011 Fiesoli viene nuovamente arrestato con l'accusa di violenza sessuale, violenza privata e maltrattamenti contro minori. Per il gip le testimonianze rese sono credibili e coerenti: violenze, vessazioni, abusi, obbligo al lavoro sui campi prima di andare a scuola. il rinvio a giudizio per Fiesoli, Goffredi e altre 22 persone. Nel giugno 2012 si aprono i lavori della Commissione d'inchiesta regionale, trasversale ma solo perché battezzata con un titolo abbastanza vago, altrimenti qualche consigliere di sinistra si sarebbe opposto. Alla luce di questi fatti viene da domandarsi come sia e sia stato possibile che un tribunale dei minori - tramite gli uffici comunali - abbia continuato per anni (e con diversi presidenti) ad affidare minori in difficoltà ad una comunità guidata da due persone condannate in via definitiva per reati a sfondo sessuale. Com'è possibile che un tribunale dei minori - un'istituzione dello Stato - abbia per anni affidato minori in difficoltà ad una comunità il cui *guru* teorizza pubblicamente, in libri e convegni, forme di famiglia *contra legem* (la cosiddetta famiglia funzionale)? Com'è possibile che, nonostante la legge preveda la durata massima degli affidi in due anni più due, gran parte dei bambini del Forteto vi siano rimasti ben oltre i quattro anni? Com'è possibile, inoltre, che nel corso quantomeno degli ultimi quindici anni non un assistente sociale si sia accorto delle anomalie - per usare un eufemismo - come, ad esempio, bambini affidati a coppie reali ma di fatto assegnati ad altre. Com'è possibile che da parte degli enti preposti non ci siano stati controlli accurati a carico di una comunità che accoglieva decine di minori in difficoltà, quando una coppia che avvia l'*iter* per un'adozione o un affido deve seguire un *iter* lungo e complesso e, successivamente, controlli periodici? Com'è possibile, infine, che le istituzioni abbiano continuato a sostenere economicamente e simbolicamente Il Forteto, nonostante le lunghe ombre che da anni gravavano su quella comunità? Com'è possibile che le istituzioni abbiano concesso un finanziamento per un progetto di scolarizzazione, nonostante sia facilmente provabile che al Forteto la maggior parte dei bambini lasciava la scuola dopo le medie? Domande la cui risposta non può che essere a dir poco inquietante. Certo è che alla base di questo scandalo c'è stata una rete di amicizie e relazioni che spesso si è trasformata in un reticolo di connivenze e di complicità politiche, sodalizi di matrice ideologica e culturale che hanno permesso il perpetuarsi di fatti come quello - sconcertante nella sua unicità - de Il Forteto: un presidente del tribunale dei minori che affida bambini e ragazzi disagiati a una comunità che incarna - seppur in maniera distorta - le sue convinzioni, tanto da spingerlo a proseguire gli affidi anche dopo una denuncia e la disposizione di una misura cautelare. Qui il garantismo non c'entra: in discussione non c'era e non c'è la decisione di scarcerare Fiesoli in attesa del giudizio, ma quella di continuare ad inviargli bambini in difficoltà, senza prendere nessuna cautela nei confronti dei minori. Che i fatti abbiano dimostrato che quella decisione era sbagliata è irrilevante: interrompere gli affidi sarebbe stato in ogni caso il provvedimento più giusto a tutela dei minori. Evidentemente lo spirito di appartenenza e la condivisione del medesimo apparato ideologico ha prevalso su tutto, perfino sulla tutela di bambini già costretti a vivere una situazione di disagio. Giudici minorili, uffici comunali, assistenti sociali, esponenti politici e sindacali: in tanti hanno avuto contatti con Il Forteto nel corso di questi decenni, in tanti sarebbe potuto sorgere almeno un dubbio. Così non è stato. In tanti non hanno visto o non hanno voluto vedere, non hanno capito o non hanno voluto capire. Oltre agli affidi, i mancati controlli, con i servizi sociali comunali, che - per stessa ammissione degli assistenti sociali - in occasione delle verifiche periodiche conferivano deleghe talmente specifiche da impedire ispezioni approfondite: controlli che peraltro venivano preannunciati alla comunità, quasi a voler dare il tempo di mettere ordine, di nascondere i panni sporchi. sporchi. Infine, esponenti politici che facevano spesso tappa al Forteto in quanto soggetto sociale ed economico rilevante, uscendone spesso - come hanno raccontato i ragazzi - con buste della spesa piene di prodotti della cooperativa. Ricordo le istituzioni che hanno continuato a finanziare la comunità e sono state in *partnership* con Il Forteto: la Regione e la stessa università, con importi anche di 670.000 euro, o ancora il sindaco cui era giunta la richiesta di incontro da parte di una maestra che aveva riscontrato anomalie nei comportamenti di un bambino del Forteto, che ottenne un appuntamento ma vi trovò Fiesoli anziché un rappresentante del Comune. Ritengo quindi sia un dovere del Parlamento attivarsi finalmente per fare piena luce su questa vicenda, figlia di un apparato ideologico tardo-sessantottino, basato sulle utopie comunitarie, sul rifiuto della società borghese e dei suoi legami, della famiglia, vista come gabbia oppressiva da cui fuggire, che ha ispirato la nascita del Forteto. Quello che preme qui è cercare di capire le ragioni di un silenzio durato quasi trent'anni e creare le condizioni e gli anticorpi perché nessuno in futuro rimanga più impigliato nella stessa ragnatela.

nei mesi scorsi la II sezione penale della corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna per dieci imputati della comunità-setta Il Forteto, dove per quasi quarant'anni più di ottanta ragazzi hanno convissuto con violenze sessuali e maltrattamenti. Nelle motivazioni della sentenza, rese pubbliche cari colleghi - nel gennaio scorso, i giudici si soffermano soprattutto sulla figura di Rodolfo Fiesoli, fondatore de Il Forteto, al quale è stata confermata dalla Corte la condanna a quindici anni e dieci mesi, nonché sulla natura dei maltrattamenti e delle violenze consumatesi nella stessa comunità. Su Fiesoli i giudizi utilizzano parole precise e crude: «Dai modi bruschi e scurrili, con uomini e donne, sempre pronto a usare le mani». il passaggio che dovrebbe farci riflettere di più è quello sui maltrattamenti e le punizioni che venivano inflitte ai minori. I maltrattamenti - si legge nelle motivazioni - «non si compendiavano esclusivamente in aggressioni fisiche o o offese, ma si applicavano vieppiù in condizioni umilianti, sminuenti, castranti tese a comprimere la psiche della vittima». Parole, quelle dei giudici, che hanno un significato ben preciso e non lasciano dubbi sulle violenze aberranti perpetrate nei confronti di bambini e ragazzi indifesi all'interno della Molti sono però gli interrogativi su come si sia potuto verificare tutto questo e su come sia potuto continuare nel tempo. Nessuno in questi anni ha sentito mai il dovere e la necessità

se facciamo riferimento al *dossier* prodotto dalla Commissione d'inchiesta della Regione Toscana, in cui si denunciavano compiacenze e coperture della politica regionale su questa vicenda. Proprio questo è uno degli aspetti sui quali la Commissione d'inchiesta dovrà fare chiarezza: accertare i fatti e le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità Il Forteto, anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte poste in essere all'interno della comunità. Anche in questa agghiacciante vicenda la volontà di nascondere la polvere sotto il tappeto ha avuto il sopravvento sulla volontà di fare chiarezza, che ha dimostrato al contrario la collega Bottici. Se non viene immediatamente adottata una strategia capace di garantire il costante monitoraggio delle strutture di accoglienza, è chiaro che questa terribile storia non ci avrà insegnato nulla. Se non mettiamo in campo una serie di iniziative volte a verificare il reale funzionamento di tutte le strutture presenti sul territorio nazionale, comprese quelle che ospitano gli immigrati, significa che non vogliamo individuare e risolvere eventuali situazioni simili a quelle del Forteto, che potrebbero essere presenti sul territorio nazionale. ben venga, quindi, la possibilità riconosciuta da questo disegno di legge alla Commissione d'inchiesta di formulare proposte circa l'adozione di nuovi strumenti di controllo sulle comunità d'alloggio presenti sul territorio nazionale. Se non faremo questo, se non procederemo in questa direzione, a pagare un prezzo carissimo sono e saranno sempre i minori e le famiglie d'origine, che subiscono sempre di più l'allontanamento frettoloso e inopportuno dei propri figli. Lo scarso rispetto per la famiglia d'origine emerge anche nel anche nel caso del Forteto e sono gli stessi giudici d'appello a rilevarlo nelle pagine delle motivazioni della sentenza nei confronti di Fiesoli: «Rigide regole di separazione dalla famiglia d'origine» - si legge - «denigrata e calunniata». Parole sulle quali, colleghi, dovremo seriamente riflettere e che testimoniano ancora un volta quanto sia necessaria e urgente una riforma complessiva e sostanziale dell'istituto dell'affido civile, volta alla tutela e al supporto della famiglia d'origine, all'incentivazione dell'affido familiare e al sensibile ridimensionamento delle strutture di accoglienza.

o meglio, è il caso estremo di una situazione che purtroppo è nazionale e rivela carenze enormi nella gestione dei minori fuori famiglia.

è che, nonostante le numerose denunce, nonostante addirittura gli arresti del protagonista, del *guru*, del santone che guidava questa comunità, a tale

un tribunale gli affidava un minore in più da violentare, da rovinare e da ridurre in stato di schiavitù. Sono cose incredibili ed è incredibile che si debba arrivare ad

che, salvo rarissimi casi, quando è andata bene hanno proposto giusto un assaggino del rendiconto di questa situazione:

organizzazione. Ci sono tribunali che non hanno agito, magistrati di altissimo rango - dal punto di vista della carriera nella magistratura - che andavano in visita in questi posti, non si accorgevano di nulla

uno spazio per cui queste cose possono avvenire, perché l'intero sistema della gestione dei minori fuori famiglia ha delle carenze enormi.

Ci sono stati casi, che io ho denunciato con una serie di interrogazioni (ovviamente senza risposta) e con conferenze stampa, che, trattandosi di minori abusati fuori famiglia, non possono riscontrare l'interesse dei grandi *media*, che si occupano d'altro. Si interessano di ciò che loro ritengono fondamentale, cioè difendere, direttamente o indirettamente, gli interessi delle grandi forze finanziarie che stanno dietro questi mezzi di informazione. Ma la realtà resta. La realtà, ad esempio, è che dal 2011 il Governo dell'epoca (ma il Governo ha una sua continuità) si era impegnato ad allestire una vera anagrafe, un vero registro dei minori fuori famiglia.

quanti sono in ogni struttura e quali sono i piani messi in atto dai tribunali e dai servizi sociali per dare una prospettiva a questi giovani, cioè il loro ritorno alle famiglie di origine, quando è possibile, oppure la loro adozione da parte di altre famiglie. Questo

cui dati sono completamente inattendibili in quanto contrastano con ciò che si può rilevare in alcuni casi andando sul posto. Faccio un esempio: quando dicono che in una provincia non c'è neanche un minore fuori famiglia e poi si scopre che ce ne sono, è evidente che questi dati sono inattendibili. Tutto quello che c'è è questo. Lì c'è lo spazio per cento strutture Naturalmente, la speranza di tutti è che le persone che hanno tenuto i criminali e inaccettabili comportamenti del Forteto siano rare; ma possono esserci, e realtà come Il Forteto possono perseverare e prosperare in molti posti nel nostro Paese,

Concludo facendo un accenno all'articolo 403 del codice civile; quella sì che sarebbe stata una legge da fare (ma purtroppo c'erano altre cose da fare). L'abbiamo sollecitata parecchie volte. L'articolo 403 del codice civile è una disposizione per cui, su decisione di una persona dei servizi sociali (non di un magistrato o di un collegio di persone, ma di una singola persona dei servizi sociali, magari supplente, magari neolaureata, magari assunta temporaneamente), un bambino può essere strappato E sapete come funziona? Non è che si porta la vicenda in tribunale e si possono opporre le proprie ragioni. No, la tipica modalità è andare a scuola quando i genitori non ci sono. I genitori hanno portato i bambini a scuola, fiduciosi che fossero al sicuro: vengono i carabinieri in uniforme, prendono questi bambini e li portano lontano da dalla loro abitazione, perché non ci sia possibilità di interazione con i loro genitori, in condizioni paragonabili ai sequestri fatti dai regimi di certi Paesi del Sudamerica (spero del passato, ma temo anche del presente). Questo è l'articolo 403 del codice civile. In alcuni casi è giusto applicarlo, perché ci sono certe famiglie che sono dei piccoli Forteto. Ma in molti casi così non è. Ci sono casi di bambini sottratti alle famiglie solo perché la casa non era abbastanza decorosa o abbastanza pulita; vengono portati lontano dai genitori e i genitori non possono sapere dove si trovano i loro bambini. Ci sono casi, testimoniati nelle mie interrogazioni, dove dei genitori, ai quali non è mai stato addebitato alcun comportamento scorretto, possono vedere i loro possono vedere i loro bambini solo mezz'ora al mese, sotto la sorveglianza dei servizi sociali, colpevoli di questo sequestro di persona. Allora, ben venga la Commissione d'inchiesta, anche se avrà la possibilità di fare solo un atto simbolico. Ma questo problema va affrontato. Spesso

oltre lo sdegno, oltre il giudizio, che sembrerebbe immediato, visto che ci sono anche condanne penali, e proprio a questo, per andare oltre, servono le Commissioni di inchiesta. Voglio essere sincera fino in fondo: io credo nelle Commissioni d'inchiesta, credo nelle inchieste parlamentari, perché il singolo

sia con le pubbliche amministrazioni, che hanno continuato a finanziare, a foraggiare cooperative che sicuramente hanno a loro disposizione soci e lavoratori degni di questo nome, ma che

ci sarà stato chi era informato e chi non lo era. Non siamo in grado ora di fare una valutazione finale su quanto successo. Ben vengano i controlli e un'inchiesta che faccia luce su ciò che non funziona nel nostro Paese perché non basta affidare.

si affidano persone e si stanziano somme da spendere. Questo evoca un altro problema che riguarda i controlli sulla gestione delle cooperative. Credo che in questo mondo ci siano esempi positivi e credo che il terzo settore e queste cooperative abbiano fatto dell'Italia

la buona pratica sia comune e diffusa in tutto il Paese e non affidata al singolo profeta di turno. Ringrazio quindi la collega. Noi voteremo favorevolmente. Sicuramente saremo parte diligente anche nell'essere parte di questa Commissione, se avrà vita,

l'avere lasciato questo segno di attenzione servirà anche nel futuro per riprendere il cammino da dove sarà stato interrotto per la fine di questa legislatura.

la comunità propriamente detta, che si riconosce nell'associazione del Forteto e dove sempre si pratica l'accoglienza dei minori in affidamento presso le cosiddette famiglie funzionali, un concetto del tutto autoctono del Forteto, che indica individui spesso tra loro in relazioni appena superficiali, ma individuati quale nucleo per la sola funzione dell'affido. Poi la cooperativa agricola, un volano consistente con un fatturato che si aggira sui 16 milioni di euro, i cui soci sono componenti della comunità. Infine, la fondazione, che si dovrebbe occupare di diffondere la filosofia del Forteto con particolare riferimento all'attività educativa - lo dico ovviamente tra virgolette - dei minori nelle scuole e all'interno della comunità Nel 2002 avvenne un fatto che credo sia utile ricordare a quest'Assemblea. Del caso del Forteto e delle sentenze che non avevano sortito effetti sulla catena di affidamenti di minori alla comunità si occupò Bruno Vespa in una puntata della

- «ci siamo occupati tante volte di minori, ma non abbiamo mai subito tante pressioni come quelle per non occuparci di questa vicenda del Forteto; pressioni quotidiane che sono avvenute con una sistematicità che francamente ci ha sconcertato. Noi ci siamo sempre occupati con grande prudenza dei minori, nessuno ha mai avuto nulla da obiettare e adesso si vorrebbe sostenere che il solo fatto di pronunciare questo nome proibito, Il Forteto, possa nuocere a questi bambini e, quindi, si vorrebbe sostenere che una trasmissione di informazione non possa dar conto di una vicenda per la quale lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Questo francamente ci pare eccessivo». A me pare invece emblematico del clima che si respirava in quegli anni e che si è continuato purtroppo a respirare fino a poco tempo fa. Mi riferisco al clima di complicità che ha avvolto tutta la vicenda del Forteto. Ma andiamo avanti. Nel giugno del 2012 il Consiglio regionale della Toscana istituì la prima Commissione di inchiesta per far luce sulla vicenda del Forteto. La Commissione concluse i lavori nel gennaio 2013, con una relazione, approvata all'unanimità, che, attraverso numerose testimonianze dai contenuti drammaticamente univoci e concordanti, ricostruì, al pari di quanto rilevato dai magistrati nella loro attività inquirente, un quadro raccapricciante. si legge che l'abuso era la prassi: le pratiche abusanti rilevate dai commissari vanno dall'abuso fisico a quello sessuale, dall'impiego del lavoro dei minori a varie pratiche di coercizione fisica e mentale, fino all'abuso psicoemotivo e affettivo, in particolare attraverso la rescissione totale dei legami con la famiglia di origine. A seguito dei lavori della Commissione fu sollevata la necessità dell'invio al Forteto di ispettori

cooperativa, purtroppo mai avvenuto. Io presentai un'interrogazione al Ministro dello sviluppo economico per avere informazioni sulla richiesta di commissariamento del Forteto avanzata dagli ispettori ministeriali. L'8 ottobre 2013 il Ministero dello sviluppo economico fece sapere, attraverso una lettera ufficiale, di aver concluso che sussistevano le condizioni per accettare la proposta di commissariamento avanzata dagli ispettori e di aver inviato il fascicolo alla direzione competente

chiese di nuovo il commissariamento del Forteto, lo scioglimento dell'associazione e della fondazione e l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta. cito alcuni passi. «È emersa chiara la responsabilità enorme del tribunale di Firenze. C'erano già state delle sentenze contro i capi del Forteto, ma il tribunale ha continuato ad affidare bambini prima all'associazione, poi a cosiddette famiglie interne a quella comunità». Ci sono state gravissime individuali, con nomi e cognomi di magistrati che hanno fatto le assegnazioni o che non hanno controllato come avrebbero dovuto, e responsabilità anche ideologiche, soprattutto nei primi anni. Responsabilità pesantissime, dunque, che coinvolgono anche i servizi sociosanitari che avevano l'obbligo di fare le verifiche e di riferire al tribunale, ma che spesso l'hanno fatto molto male. La Commissione regionale ha esplicitamente messo sotto accusa anche la politica locale, in particolare il centrosinistra, che - cito ancora testualmente - avrebbe agito «superficialmente, con molti passaggi al Forteto anche di personaggi importanti che hanno contribuito ad accreditare una immagine idilliaca di quella esperienza». Ci sono, insomma, tutti gli estremi per approvare e mettere immediatamente al lavoro questa Commissione d'inchiesta parlamentare, anche se la legislatura è vicina al suo termine. Ogni giorno sarà utile per fare finalmente luce su questo che è, a mio parere, uno scandalo nazionale. Lo dobbiamo soprattutto ai bambini vittime del Forteto, ma lo dobbiamo anche alla nostra coscienza di parlamentari. È chiaro che ci sono state immani complicità politiche in questa oscura vicenda; complicità di una vecchia sinistra ideologica, accecata dal comunitarismo anni Settanta, che vedeva nel rifiuto dell'istituto familiare e nella collettivizzazione di beni e lavoro l'affermazione di un nuovo modello di socialità. Sulla base di questo *totem* quella sinistra ideologica ha assecondato, magnificato, giustificato, accreditato e anche finanziato con fondi pubblici il delirio privato per il quale il capo carismatico del Forteto e i suoi complici accoglievano in affidamento minori in difficoltà per sottoporli a ogni tipo di vessazione e di abuso fisico, emotivo, sessuale, affettivo e psicologico. E allora: anche noi, come la senatrice Bottici che ringrazio per questa iniziativa e per la tenacia con cui l'ha portata avanti - vogliamo che sia fatta piena luce in Parlamento e si attivi una Commissione d'inchiesta sulla vicenda del Forteto e sul ruolo che la politica ha avuto in questa drammatica vicenda andata avanti per trent'anni. La giustizia dei magistrati farà il suo corso; per quella politica ci batteremo fino in fondo, affinché ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Grazie, Presidente. arriva finalmente in approvazione il provvedimento sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti della comunità Il Forteto, che noi abbiamo sempre ritenuto urgente; invece, troppo tergiversato, soprattutto alla luce della gravità dei fatti. I massimi esponenti e fondatori della comunità, che accoglieva minorenni, sono stati in più occasioni condannati - condannati! - per abusi, maltrattamenti,

le condanne e nonostante, addirittura, una sentenza della Corte di Strasburgo, che ha condannato l'Italia a un risarcimento, all'epoca, di 200 milioni di lire, il tribunale dei minori di Firenze ha continuato per decenni ad affidare bambini e adolescenti alla comunità, allontanandoli dalle famiglie in modo irrecuperabile e contribuendo a sottoporli a violenze fisiche e psicologiche gravissime. Resta da capire come mai nessuno degli attori coinvolti e responsabili (servizi sociali, Regione, servizio sanitario) sia stato in grado di tutelare i minori da un contesto che avrebbe quantomeno dovuto fare emergere seri dubbi, date le continue condanne di Fiesoli; autorità pubbliche, quindi, che sono venute meno ai loro compiti istituzionali, contribuendo ad affidare bambini e adolescenti a tale luogo degli orrori. Le ricostruzioni ci raccontano di un crimine perpetuato sotto l'egida delle istituzioni, con una colpa diluita nella generalità del sistema, in modo che fosse quasi impossibile da individuare. Vorrei ricordare che anche durante le indagini della Commissione di inchiesta della Regione Toscana vi è stato un continuo scaricare le responsabilità e barricarsi dietro le affermazioni: non mi competeva, era competenza di altri. quindi, che uno degli scopi principali della Commissione di inchiesta parlamentare dovrà essere quello di venire a capo di tali processi, di come tutto questo sia potuto accadere, contribuendo alla definitiva emersione della verità su quanto successo al Forteto,

Ricordo infatti come gli affidamenti di minori al Forteto risultano essersi interrotti solo nel 2012 a causa di un nuovo, ulteriore, arresto di Fiesoli. Nel processo che ne è seguito il pubblico ministero Ornella Galeotti ha affermato che per alcuni decenni in Toscana si è verificato un fenomeno rispetto al quale le leggi dello Stato hanno subìto una sospensione.

per avallare l'interpretazione di una sentenza di condanna chiarissima come una pronuncia di tipo politico. Ci si è barricati in molti casi dietro a questo proprio per continuare a perpetuare gli affidamenti. In questo alone di consenso è subentrata una *routine* che ha determinato l'omissività nel monitoraggio e nei controlli, nei doveri istituzionali, nonché l'assenza di qualsiasi forma di approfondimento e l'abbandono anche di un rigore serio e scientifico che non avrebbe dovuto accreditare forme di affidamento praticamente fuori da ogni logica. necessario che la Commissione accerti la verità e che sia preso ogni provvedimento affinché tutto ciò non capiti nuovamente, senza ovviamente cadere nella tentazione di accusare genericamente i servizi, o i servizi o i servizi sociali in generale, ma individuandone i meccanismi sbagliati e le responsabilità, l'incapacità di comprendere e di discernere discernere di tutti i sistemi di controllo. Certamente la Commissione avrà questi compiti molto precisi.

produttivi per fare in modo che la Commissione sia subito operativa e possa svolgere il proprio lavoro. Per tutti questi motivi

Lo dobbiamo a tutte le vittime della comunità Il Forteto, sperando che questa Commissione possa accertare finalmente la verità e le responsabilità per impedire che altri casi del genere possano verificarsi nel nostro Paese.

nella circostanza delle dichiarazioni di voto a favore del provvedimento che inaspriva le pene e argomentava ulteriormente casi di illecito operati dai custodi della giustizia (siano essi magistrati, cancellieri, avvocati), la corruzione in atti giudiziari e fatti consimili, concludevo l'intervento di allora con una famosissima citazione tratta dalla VI Satira di Giovenale che oggi torna di estrema attualità e riparto da quella: «*Quis custodiet ipsos custodes? Cauta est et ab illis incipit uxor».* Chi sorveglierà i sorveglianti? La moglie astuta La satira riguardava un attacco feroce al malcostume delle donne romane di allora, siano esse ricche o povere, nobili o plebee, e ha in questo contesto un riferimento alla tragica attualità di questa vicenda. Cioè, gli stessi organi di sorveglianza, anche quelli della giurisdizione, in un percorso quasi quarantennale, hanno consentito, per compiacenze, ignoranza, indiligenza, forse connivenze di varia natura che avvenisse questo scempio del diritto questa tutela dei deboli, questa nobile missione di tutelare i minori minacciati da angherie, da abusi sessuali e quant'altro, invece che essere causa di salvazione, fosse circostanza circostanza nelle quali questi gravi fatti venivano reiterati e ripetuti. Il primo episodio di arresto del responsabile di questa comunità risale nientemeno che al 1978, quando il giudice Carlo Casini (che io ebbi modo di conoscere come deputato europeo molti anni dopo) lo incriminò di reati sessuali. Egli viene incarcerato dopo poco tempo dalla prima carcerazione, lascia il carcere per tornare alla comunità Il Forteto; lo stesso giorno gli viene affidato, dal tribunale per i minorenni, il primo bambino Down. E il Presidente del tribunale di allora, grande amico di Don Milani, afferma (e cito dalla relazione le frasi del provvedimento) di non credere nell'indagine del giudice Casini e di ritenere Il Forteto una comunità accogliente e idonea. Nel 1982 questa comunità allarga i confini, anche patrimoniali, della propria realtà. Acquista una proprietà di 500 ettari intorno a Firenze, si trasferisce in questo luogo ameno, sviluppa, in tempi più recenti, un fatturato dai 18 ai 20 milioni di euro all'anno

Nel 1997 il Fiesoli risulta, però, ancora capo della comunità nonostante questo increscioso precedente. Nel 1998 abbiamo un caso che raccoglie l'attenzione della Corte di giustizia europea, che nel 2000 condanna lo Stato italiano al pagamento di 200 milioni di euro per danni morali.

quelle della giurisdizione, quelle dei territori, quelle dello Stato (sia la Regione Toscana che il Ministero dello sviluppo economico) hanno aperto delle azioni ispettive con esiti evidentemente non soddisfacenti. in questi quasi quarant'anni si è lasciato che questo scempio si perpetrasse. Quindi, ben venga, finalmente, da parte dell'organo legislativo,

e sulle circostanze, quasi inspiegabili, per cui c'è stata questa connivenza e questa incapacità di riconoscere gli illeciti e di interrompere questo scempio, ma che possa soprattutto ricavare, da queste esperienze e dalla conoscenza di questi fatti, utili argomenti, tracce, aspetti di funzionale applicazione di condotte che possano in futuro impedire il ripetersi di fatti del genere. Ci auguriamo davvero che la Commissione possa svolgere il suo compito e lasciare alle istituzioni della Repubblica dei segnali e degli indirizzi che possano consentirci di non dover ripercorrere questa incresciosa strada. *(Applausi Signor Presidente, era l'11 luglio del 2013 quando presentavamo la prima interrogazione in

le ragioni per cui la comunità, anzi la cooperativa Il Forteto, anche a seguito della condanna di Fiesoli per abusi sessuali e maltrattamenti, continuasse a ricevere in affidamento dei minori, anche perché quello che stava accadendo al Forteto poteva verificarsi altrove. Ebbene, il disegno di legge è del

anche questo Parlamento si è svegliato. Poi ci meravigliamo che le istituzioni locali non si siano svegliate in tempo, quando anche il Parlamento ha dormito, perché potevamo intervenire prima. Non

come Capigruppo, a mettervi d'accordo con gli altri Capigruppo alla Camera per far sì che l'*iter* alla Camera dei deputati sia veloce, quindi convocando subito i componenti per stabilire l'ordine ed il calendario dei lavori. Mi auguro anche, visto che oggi mi sembra che tutto il Parlamento si sia svegliato,

stressando voi e la Conferenza dei Capigruppo), che c'è un'urgenza. Il nostro voto sarà favorevole. Come membro della Commissione, che mi auguro si istituisca presto, presto, porterò questo fascicolo che in questi anni mi sono studiata, perché quando si parla bisogna leggere, bisogna comprendere comprendere quello che accade. Vi ricordo che nel 2005-2006 il Fiesoli ha fatto un percorso educativo con le scuole elementari, medie e superiori in accordo con l'Università di Firenze e alcuni soggetti coinvolti

Grazie, Presidente.

lo scandalo inaccettabile avvenuto nell'ambito di quella cooperativa. Quello che è accaduto è un racconto da lager, da film degli orrori,

Quella comunità ricevette un finanziamento, dal 1996 al 2010, di oltre 1,2 milioni di euro dalla Regione Toscana, nonché fondi dalla Comunità europea. Già trent'anni prima si sperimentava omosessualità, pedofilia e zoofilia: tutto quello che era la negazione della natura, come se regnasse un'anarchia morale. Si sarebbe potuto fermare tutto questo un anno dopo l'apertura, quando un magistrato arrestò il fondatore Roberto Fiesoli per violenza sessuale. Ma non servì. Venne scarcerato e ci fu una presa di posizione politica e fortemente ideologica della comunità che lo sosteneva, con l'affermazione che le denunce di violenza erano solo frutto di malelingue. Fiesoli si faceva chiamare «il profeta». Riuscì - non si sa bene come, vista la scarsa credibilità che avrebbe dovuto avere - a organizzare conferenze. Antonio Di Pietro tenne persino una conferenza contro la pedofilia al Forteto; lì passarono Livia Turco, Rosy Bindi e Fassino, ma nessuno si accorse di quanto succedeva e delle denunce sporte. Addirittura, nel febbraio 2010, il Gruppo del Partito Democratico presentò al Senato un libro scritto da Fiesoli. Vorrei citare una parte della motivazione della sentenza della seconda sezione penale della corte d'appello di Firenze, quando ha condannato a quindici anni questo mostro: «Dai modi bruschi e scurrili, con uomini e donne, sempre pronto a usare le mani e abbassarsi i pantaloni mostrando il proprio membro, non si sa bene per quale fine propedeutico o educativo». sui maltrattamenti: «Non si compendiavano esclusivamente in aggressioni fisiche o offese, ma si applicavano vieppiù in condizioni umilianti, sminuenti, castranti tese a comprimere la psiche della vittima». Mi chiedo dunque come mai - ed è la domanda che molti ci poniamo in quest'Aula e fuori - i giudici minorili, gli assistenti sociali e i servizi sociali continuavano ad affidare i minori

Non è chiaro nemmeno come mai la Regione Toscana abbia voluto escludere dal Salone del libro di Torino, conclusosi pochi giorni fa, il libro inchiesta sulle vicende del Forteto, intitolato come d'altronde si evince dagli atti del Consiglio regionale della Toscana, quando fu respinta la proposta di risoluzione, sottoscritta da vari Gruppi, con cui si presentazione di questo libro a tale Salone. Fiesoli è stato condannato in primo grado per questi fatti gravissimi nel 1981 (ma già nel 1980 un consigliere regionale aveva denunciato la situazione di violenza), ma un giudice molto famoso fece poi dimenticare il verdetto e tutto rimase come prima. Dal 1985 ci fu un dominio incontrastato di Fiesoli al Forteto.

minimo di giustizia alle vittime di violenza, ammettendo quello che era successo in tutti questi anni. Spero che emergano tutte le responsabilità, anche di alcuni dirigenti della cooperativa, che deve comunque continuare un'attività per questo che il Governo emani un decreto *ad hoc*. Sono molto rammaricata del ritardo con cui si dà il via libera alla Commissione d'inchiesta, nonostante le ripetute richieste in Consiglio di Presidenza. Spero veramente che ci sia un rapido esame del testo deputati, per poter cominciare a lavorare al più presto, altrimenti questi ulteriori ritardi farebbero pensare maliziosamente, come diceva il nostro Andreotti.

oggi l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto. In Commissione Giustizia abbiamo esaminato il testo con cura e lo abbiamo arricchito in alcune sue parti. I richiamati, già esposti dalla relatrice e via via supportati da diversi interventi sono gravissimi, per alcuni versi terribili: bambini allontanati dalle famiglie d'origine, bambini sottoposti ad abusi fisici, sessuali e psicologici. Come mai? Perché è successo? Quali responsabilità ci sono state? Quali controlli sono andati a vuoto? Perché non si è colta subito la drammaticità della situazione, dopo la prima condanna dei fondatori? responsabilità diverse e ripetute, ma che non possono più andare a vuoto. La magistratura penale ha agito, ci sono state due commissioni di inchiesta a livello della Regione Toscana. indaghi con i poteri tipici di una Commissione d'inchiesta, non si guardi in faccia a nessuno e si agisca con rigore e serietà, senza richiami strumentali alle culture politiche o alle nostre rispettive appartenenze.

il compito di formulare proposte in ordine: *a)* all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; *b)* al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori». I minori meritano il meglio del Paese, soprattutto quando sono in difficoltà, sia di tipo sociale che familiare. Si vadano a verificare le varie responsabilità e si gettino le basi per sostenere le comunità oneste, che nei territori lavorano in silenzio, con professionalità e amore, tra mille difficoltà e ostacoli. Allo stesso tempo siamo chiamati a rimuovere tutte le collusioni e tutte le protezioni e complicità, che proteggono i vari Forteto ancora presenti in Italia. Colleghi, daremo il nostro contributo con impegno e passione, insieme a tutti i i parlamentari pronti a fare un lavoro d'inchiesta, come la nostra coscienza detta e la Costituzione comanda. Il Partito Democratico voterà a favore della costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti della

di inserire all'ordine del giorno della seduta in corso la discussione della relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (Doc. XVI-*bis,* n*.* 11). Sulla predetta proposta può parlare un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti. La deliberazione è adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti e avrà luogo mediante procedimento elettronico. Poiché nessuno chiede di intervenire, indìco la

Signor Presidente, la relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, approvata lo scorso 10 maggio, giunge al termine di un'approfondita riflessione sullo stato del regionalismo e, più in generale, sull'assetto degli enti territoriali del nostro Paese. Si tratta di una riflessione che tiene conto delle principali criticità nel sistema di raccordo tra Stato ed enti territoriali, nell'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale e nel processo di riordino degli enti locali, secondo le indicazioni emerse nel corso delle indagini conoscitive concluse dalla Commissione, in particolare quella sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al sistema delle Conferenze; nonché quella sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. Prima di entrare nel merito dei contenuti della relazione, permettetemi di rivolgere un ringraziamento al presidente, onorevole D'Alia, per la modalità con cui ha condotto i lavori della Commissione, e a tutti i colleghi, che hanno contribuito alla stesura di un documento ampiamente condiviso, secondo una logica *bipartisan* tesa ad evidenziare criticità e a proporre soluzioni concrete nell'esclusivo interesse del Paese. Richiamo solo due numeri, che fanno comprendere l'impegno profuso dalla Commissione: considerate congiuntamente le due indagini conoscitive e l'ulteriore breve procedura informativa condotta durante l'esame della relazione, la Commissione ha svolto ben 49 sedute e audito oltre cento personalità, Un ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno contribuito ai lavori, a partire proprio dai numerosi rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore, che hanno indubbiamente arricchito i lavori della Commissione La Commissione si è altresì avvalsa della proficua collaborazione di consulenti, svolta a titolo gratuito. Infine, un apprezzamento e un sentito ringraziamento va alle due amministrazioni di Camera e Senato, che hanno fortemente sostenuto l'attività della Commissione, mettendo a disposizione personale di qualità in un'ottica di messa a sistema delle rispettive risorse. In particolare, insieme agli uffici della Commissione, voglio ringraziare i funzionari, la dottoressa Martuscelli e il dottor Fucito. Entrando nel merito, la relazione enuclea una serie di indicazioni concrete per la ridefinizione volte a completare il quadro istituzionale delineato dalla riforma costituzionale del 2001. Il primo tema affrontato riguarda l'esigenza di procedere all'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali. I soggetti auditi hanno, infatti, convenuto sulla necessità di riconoscere una sede parlamentare di dibattito e confronto sulle questioni relative agli enti territoriali, individuata nella Commissione parlamentare secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al riguardo, ricordo che l'articolo 11 demanda ai Regolamenti parlamentari l'integrazione della Commissione con rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali e stabilisce una particolare valenza procedimentale al parere reso dalla Commissione, se riferito a disposizioni di legge che incidano sulle materie assegnate alla competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) o sull'autonomia finanziaria delle autonomie (articolo 119 della Costituzione). Nel caso in cui la Commissione di merito non si adegui al parere, «sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea L'integrazione della Commissione era delineata come una soluzione-ponte in attesa di una più ampia riforma costituzionale che trasformasse il Senato in una Camera delle autonomie. Con la mancata entrata in vigore sia della riforma costituzionale del 2006, sia di quella del 2016, tale soluzione non si può considerare neanche più transitoria; piuttosto, essa costituisce l'unica forma di raccordo fra Stato ed autonomie territoriali prevista a livello costituzionale, in un assetto che può oramai ritenersi consolidato. Il ritardo nell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha costituito per il Parlamento una sostanziale rinuncia

11, lungi dal costituire una soluzione anacronistica, risulta dunque quanto mai urgente nella fase attuale, per superare l'*impasse* dovuta all'assenza di uno spazio parlamentare per la composizione degli interessi degli enti costitutivi della Repubblica. Occorre porre rimedio all'assenza di una sede istituzionale e trasparente dove le istanze provenienti dai territori possano confrontarsi con lo Stato centrale al fine di elaborare soluzioni comuni e condivise. La partecipazione delle autonomie territoriali al procedimento legislativo consentirebbe, per così dire, di anticipare a monte il confronto fra Stato ed enti

«perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi - anche solo nei limiti di quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». L'urgenza di procedere all'integrazione della Commissione si lega anche alla recente sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale. Mutando il proprio precedente orientamento, la Corte ha esteso l'applicabilità del principio di leale collaborazione all'ambito del procedimento legislativo: nei casi in cui «il legislatore delegato si accinge a riformare

il quadro del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

attivazione delle sinergie tra la Commissione parlamentare e i rappresentanti di Regioni ed enti locali, tanto per l'urgenza con cui si impongono le questioni relative all'assetto ordinamentale e finanziario degli enti territoriali, quanto per l'opportunità di porre le basi, anche metodologiche, del lavoro della futura Commissione in composizione integrata. Altro tema importante della relazione, peraltro connesso con il precedente, riguarda l'esigenza di una razionalizzazione del sistema delle Conferenze. Fra le principali criticità delle Conferenze intergovernative, dalle audizioni è emersa l'eterogeneità delle materie all'ordine del giorno e la conseguente necessità necessità di concentrare l'attività sugli ambiti propri del confronto fra Governo nazionale ed esecutivi degli enti territoriali. Si segnala inoltre l'opportunità di sostituire le tre Conferenze con una Conferenza unica, articolata in una sede plenaria e in due distinte sezioni (regionale e locale). Nell'ambito delle Conferenze, dovrebbe essere poi favorita una maggiore bilateralità,

l'assenza di una vera sede politica in cui il Governo nazionale e gli esecutivi territoriali si confrontino sulle grandi scelte strategiche per il Paese. Si suggerisce, quindi, l'istituzione di una Conferenza degli esecutivi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con il compito di delineare un'agenda politica condivisa Il terzo tema affrontato dalla relazione riguarda le Regioni a Statuto speciale. Il lavoro della Commissione si è articolato su due versanti: la revisione degli Statuti speciali e l'attuazione delle norme statutarie. Si tratta di due aspetti fra loro connessi: per un verso, infatti, l'esito non confermativo del *referendum* costituzionale

attenzione è stata dedicata alla questione dell'ordinamento finanziario delle Regioni ad autonomia speciale. L'ultimo tema affrontato dalla relazione è quello del riordino degli enti di area vasta: Province e Città metropolitane. All'indomani del *referendum* costituzionale, si è avviato un dibattito sulle possibili conseguenze della mancata entrata in vigore della riforma della Costituzione sulla legge n. 56 del 2014, con cui si è operato il riordino. In proposito, rimane immutata la collocazione nell'ordinamento delle Province, che continuano a essere enti costitutivi della Repubblica assieme allo Stato, le Regioni, Regioni, le Città metropolitane e i Comuni e a vantare una propria autonomia anche in termini finanziari. Ed è proprio alla luce della posizione di equiparazione agli altri enti territoriali delle Province che deve essere rapportata ogni ipotesi di intervento ulteriore che incida sugli enti di area vasta. La relazione ritiene auspicabile che ogni riflessione in non possa non tener conto delle trasformazioni a livello territoriale nel frattempo intervenute, e in particolare della rilevante attività legislativa posta in essere dalle Regioni in attuazione della legge n. 56 (peraltro esaminata in dettaglio da un'analisi del Servizio studi del Senato). Le Regioni hanno proceduto, infatti, ad una complessiva ed estremamente assetti degli enti locali, che si è accompagnata a una riorganizzazione delle strutture amministrative regionali e degli enti di area vasta (che ha riguardato anche procedure di mobilità di personale, ormai definite). Si tratta di un processo, in fase molto avanzata, che sembrerebbe opportuno non rimettere completamente in discussione, al fine di non introdurre elementi di incertezza in ordine all'esercizio delle funzioni appena riordinate e all'erogazione dei servizi ai cittadini. Più che ad una rivisitazione della legge n. 56, l'attenzione dovrebbe essere posta in particolare su alcune misure che, come sostenuto anche dalla Corte dei Conti in audizione, hanno inciso significativamente sull'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti di area vasta e che fondavano la loro legittimità proprio nella prospettiva della riforma costituzionale. È stata l'esiguità delle risorse, risultante dalla contestualità del taglio dei trasferimenti statali e del ritardo nell'attuazione del federalismo fiscale, che ha fatto sì che non fosse sempre pienamente assicurata la corrispondenza fra funzioni affidate

In particolare, mi voglio riferire, per esempio, alla necessità di superare i contenziosi ancora diffusi e presenti che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni. La Commissione per le questioni regionali ha riconosciuto che continuano a essere valide in alcuni ambiti

è un limite del nostro ordinamento - un luogo dove intervenire nella fase legislativa già per conciliare diverse esigenze tra Stato e poteri locali. qui nasce la necessità di mettere mano alle norme per cercare una sempre maggiore armonia tra lo Stato e le Regioni. Stato e le Regioni. Il documento appare però ancora troppo generico perché si possa prendere una posizione chiara e condivisa da parte della nostra forza politica e, presumo, anche delle altre. altre. Nonostante contenga degli elementi positivi, contiene anche degli aspetti che fanno venire dubbi sul futuro assenso che può essere dato o meno a una riforma che preveda una diversa funzione e composizione innanzitutto della Commissione per le questioni regionali. Stiamo parlando dell'ipotesi di allargare questa Commissione a rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. È un'indicazione che ci perviene dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che, al suo articolo 11,

fare alcuni esempi che inducono perplessità e prudenza nel dare assenso alla relazione. Ad esempio, l'ipotesi di allargamento a rappresentanti degli enti locali della Commissione comporterebbe ovviamente la presenza di rappresentanti delle Regioni. E fin qui nessuna obiezione.

cui delle persone nominate non da cittadini, ma da loro colleghi, ossia consiglieri comunali, si troverebbero addirittura, in un'elezione indiretta di secondo grado, a dover nominare dei componenti di una Commissione parlamentare. Quindi, avremmo componenti di una Commissione parlamentare eletti da persone che non sono elette dal popolo. Questo, soprattutto per chi fa parte del Movimento 5 Stelle, è una cosa abbastanza discutibile e bizzarra. Per questo motivo, bisognerà valutare quali saranno i testi proposti per operare l'eventuale modifica

che dovrebbero essere approvati non più a maggioranza dei presenti dalle due Camere, ma a maggioranza assoluta qualora la maggioranza della Commissione per le questioni regionali lo chiedesse.

una terza Camera. Io credo che vada assolutamente evitata un'ipotesi del genere, cercando di limitare il numero dei componenti. C'è anche da dire che la legge costituzionale del 2001 attribuisce ai Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la possibilità di prevedere una partecipazione allargata. Quindi, si dovrebbe procedere con una modifica

di fatto non dà alcuna precisa soluzione al problema del coinvolgimento delle Regioni nell'attività legislativa statale. La posizione del

Grazie, Presidente.

Proprio questo elemento, che è stato suggerito e posto con evidenza nella riforma del Titolo V del 2001, è lì a dimostrare quanto tempo sia passato da quell'atto ai giorni nostri. nostri. La mancata riforma costituzionale mette ancora più in evidenza l'obbligo di dare piena attuazione

Tra l'altro, questo passaggio prevede in sé un atto semplice, cioè l'attivazione dei Regolamenti parlamentari,

il Senato pongano mano al tema dei Regolamenti parlamentari e, in tale circostanza, diano piena attuazione alla composizione della Commissione.

Il rapporto che viene individuato nella risoluzione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali è un tema centrale: quel rapporto è il fulcro nevralgico della Repubblica. È chiaro che, se quell'elemento si inceppa, tutto rischia di essere molto più difficile, sia sul fronte della disarticolazione, sia nella capacità di dare risposte alle questioni che man mano si pongono.

il tema delle revisioni e delle attuazioni delle specialità è stato discusso, proprio in quest'Aula, ai tempi della riforma e indubbiamente richiede

derivano tanto dalla riforma strutturale, quanto dalle condizioni in cui i bilanci degli enti locali, a causa della crisi e dell'alto debito, si trovano.

indubbiamente autoapplicativa per una parte su cui, pur dichiarando il nostro parere favorevole, ci rimettiamo alla volontà del Parlamento; per l'altra parte di sollecitazione al Governo,

Signor Presidente, colleghi senatori, la relazione al nostro esame può essere considerata un testo di transizione, come è stato già evidenziato dal senatore Cotti, e per questo ha delle volute incompiutezze e delle indefinitezze, frutto anche del fatto che questa è la prima relazione che viene dopo il fallimento

forse il più importante è proprio quello che riguarda la revisione del rapporto tra autonomie e Stato. Signor Presidente, lasciando da parte le problematiche dei Comuni, che molto spesso stanno diventando degli uffici esattoriali dello Stato, e limitandoci agli aspetti che sono stati presi in considerazione dalla relazione, noi ci troviamo in una situazione nella quale - per procedere con l'accetta e certamente per stigmatizzare alcune posizioni - abbiamo delle Province che dovevano essere superate e che, come è stato giustamente rilevato dalla relazione, rimangono in Costituzione tra gli organi fondamentali dello Stato. Queste Province sono diventate organi di secondo grado, sono state esautorate di gran parte delle loro risorse ma non delle loro funzioni, con il risultato che quelli che erano compiti primari, come la manutenzione delle strade e delle scuole, sono compiti sempre più dimenticati.

le Città metropolitane, anch'esse citate in Costituzione, restano - se ne osserviamo il funzionamento - una sorta di mistero Le Città metropolitane avrebbero dovuto rappresentare il connubio tra i grandi centri e la cinta

che avrebbero dovuto determinare da una parte dei risparmi e, dall'altra, un miglioramento dei servizi. Nella loro attuazione, le Città metropolitane di tutto ciò! Sono, nel migliore dei casi, delle super Province che vengono affidate al sindaco del capoluogo, il quale, tra l'altro,

coloro i quali lo hanno sfiduciato mentre lui rimane in carica, perché in quasi tutte le città metropolitane la funzione del Presidente è una funzione stabile. Evidentemente, con questi presupposti è difficile pensare a un organismo che possa in qualche modo avere una ragione e una efficienza. La situazione è

non è riuscita ad essere quell'organo dotato di responsabilità legislativa e finanziaria che rispondesse in qualche misura ai cittadini. Il centrodestra ci ha provato nella scorsa legislatura. Il federalismo fiscale era il tentativo di incarnare questo ideale. Siamo rimasti a metà strada, sicché oggi noi ci ritroviamo con un ente fondamentale situato in una sorta di limbo, sospeso tra un passato che è bene dimenticare ed un futuro che non si è riuscito ancora a inverare. Signor Presidente, lungo questa strada ci si presenta nei prossimi mesi, anche politicamente, una grande occasione. Noi sappiamo che in autunno si svolgeranno *referendum* sull'autonomia in Lombardia Veneto. Questa occasione, che poi è maturata e anche dal punto di vista costituzionale ha determinato un capitolo importante nello nello svolgimento della vita materiale delle nostre istituzioni, può essere interpretata in due modi diversi: di due Regioni, ovvero come la grande occasione per ripensare il rapporto tra Stato e Regioni, facendola fare diventare una grande occasione nazionale. Signor Presidente, se noi interpretassimo correttamente il concetto di autonomia, dovremmo arrivare alla conclusione questo è il metro che potrebbe guidare il rapporto Stato-Regione non soltanto per Veneto e Lombardia, ma per tutte le Regioni italiane. E alla luce di questa impostazione potremmo riaprire il dibattito sulla specialità, che pure è stato citato nella relazione, evidenziando come il superamento di questa specialità - d'altra parte alcuni elementi ci sono stati forniti dalla senatrice Orrù in questo senso - in questo senso - può avvenire non attraverso l'abrogazione, ma attraverso il riconoscimento del fatto che il rapporto tra ogni singola Regione e lo Stato dovrebbe essere speciale, se in qualche modo governato

dunque l'autonomia dovrebbe essere un concetto a geometria variabile, perché quello di cui ha bisogno la Lombardia è diverso da quello di cui ha bisogno la Sicilia e quello di cui ha bisogno il Nord è diverso da quello di cui ha bisogno il

potrebbe essere alla base di una profonda riforma. D'altra parte queste non sono idee originali: si tratta di considerazioni già emerse nel dibattito costituente. Basti pensare alla riflessione di quegli anni di un politico come come don Sturzo per comprendere come, tornando a quella radice, noi potremmo fare un passo in avanti. In conclusione, signor Presidente, il nostro voto sarà voto sarà favorevole ed è un voto di incoraggiamento; è il voto di chi ritiene che si sia fatto lo sforzo di tematizzare la transizione ma che ora sia necessario andare avanti e non mettere assolutamente sotto il tappeto un tema che è fondamentale per la vita del nostro Paese e del nostro Stato per i prossimi decenni.

Signor Presidente, noi ci saremmo aspettati una presa d'atto più coscienziosa e più forte, ovviamente da parte della politica che sostiene la maggioranza, dei guasti generati

invece trovati di fronte prima alla legge Delrio, con tutti i guasti che ne derivano, e poi di fronte alla riforma costituzionale, di cui conosciamo bene i devastanti risultati. Nella relazione troviamo delle affermazioni rispetto alle quali non possiamo che essere contrari, a partire dalle considerazioni che nella relazione vengono fatte riguardo al riordino degli enti di area vasta, perché non si può non prendere atto del fatto che i guasti causati dalla legge Delrio devono essere superati di slancio, andando semplicemente a rimuovere la modifica di un assetto che, prima ancora di essere costituzionale, è stato ordinamentale. Hanno cominciato a smontare la casa dalle fondamenta, non facendo attenzione al fatto che il tetto poi è rimasto pericolante, nel momento in cui la stessa casa è rimasta pericolosamente in bilico. Oggi ci troviamo con le Province che continuano a esistere e con la sovrapposizione degli enti di area vasta, con la definizione delle città metropolitane che non troveranno mai una loro compiuta attuazione, in un sistema che sta invece depredando gli enti locali, nel caso specifico le Province, delle risorse che dovrebbero essere alla base di qualsiasi politica amministrativa.

che non necessitano di una riforma costituzionale. In essa si parla di Conferenze unificate e di integrare i rapporti che oggi già esistono con la Conferenza Stato-Regioni: tutte misure insufficienti.

Grazie, l'approvazione del passaggio del Comune di Sappada da una Regione all'altra, e guarda caso da una Regione a Statuto ordinario a una a Statuto speciale. In questa relazione è dedicato pochissimo spazio al rapporto tra le Regioni a statuto ordinario e quelle a Statuto speciale, quando le disequazioni ormai sono evidenti, in un Paese che non ha trovato, attraverso il regionalismo differenziato, l'opportunità di una maggiore unità.

tenendo conto delle indicazioni in essa contenute. Avremmo voluto che nella relazione si fosse parlato diffusamente della voglia di libertà e autonomia che contraddistingue i cittadini lombardi e veneti, che il prossimo 22 ottobre saranno chiamati a esprimersi, con un *referendum* libero, sul loro diritto a chiedere al governo regionale di portare la loro Regione ad avere più autonomia. È una rivendicazione di principio che, nel momento in cui sarà attuata in Lombardia e in Veneto, potrà essere seguita in altre Regioni italiane, perché questa è la differenza che sta tra noi e voi: chiamare il popolo a esprimersi per noi è un valore aggiunto, mentre per voi è un problema da cui uscire.

non vuole consentire che un Comune passi da una Regione a statuto ordinario ad una a Statuto speciale. Altrimenti - quello che non viene detto, ma è scritto tra le righe - quanti altri Comuni seguirebbero il suo esempio?

Voteremo contro questa relazione, perché è ipocrita nel contenuto e vuota nelle prospettive che offre. Le uniche serie prospettive che possono essere date al Paese per uscire dalla crisi, che ancor prima che economica è politica, sono quelle di riconoscere i livelli di autonomia a cui i cittadini di tutte le Regioni, oltre a quelli lombardi e veneti, hanno diritto ad ambire e aspirare. Con questi presupposti voteremo contro la relazione e invitiamo il Governo ad una seria riflessione.

Signor Presidente, innanzitutto voglio evidenziare il significativo lavoro svolto dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali in ordine ai rapporti fra Stato ed enti territoriali. Si tratta di un lavoro complesso, articolato, che ha fra l'altro previsto l'audizione dei soggetti interessati, che credo sia sinonimo della vitalità della nostra democrazia rappresentativa. Con la relazione della Commissione, approvata il 10 maggio 2017, si intende così portare a compimento il percorso intrapreso negli ultimi due anni con lo svolgimento di due indagini conoscitive sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle Conferenze», e sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. A parere del nostro Gruppo è opportuno evidenziare in questa sede alcuni temi di particolare rilievo. Va sottolineata innanzitutto la mancata attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Da questo punto di vista l'attuazione del citato articolo risulta dunque quanto mai urgente, per superare la complessa situazione causata dall'assenza di uno spazio parlamentare per la composizione degli interessi degli enti costitutivi della Repubblica. Sotto questo profilo, infatti, emerge dalla relazione che la Commissione parlamentare per le questioni regionali in composizione integrata potrebbe avere un ruolo fondamentale per la prevenzione del conflitto costituzionale tra Stato e Regioni. Si ricorda a tale proposito che attualmente l'unico organo in grado di assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di governo è rappresentato dal sistema delle Conferenze (Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città e autonomie locali e Conferenza unificata), che sono sicuramente un luogo di concertazione degli esecutivi dei vari enti territoriali, ma non certamente la sede più adatta qualora si intenda intervenire sul piano della funzione legislativa. La relazione fa poi emergere una possibile soluzione a questa problematica, attribuendo alla Commissione in composizione integrata potere consultivo su tutti i progetti di legge di interesse per gli enti territoriali, mantenendo dunque una competenza inalterata rispetto a quella della attuale Commissione parlamentare per le questioni regionali. In tal modo la Commissione in composizione integrata potrebbe pronunciarsi su materie di fondamentale importanza per il governo territoriale, come l'ordinamento degli enti locali, che risulta attribuito alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della nostra Costituzione. Sul fronte poi della revisione e dell'attuazione degli Statuti ad autonomia speciale la relazione ci consegna senza dubbio un campo di future attività, che mirano nella sostanza a determinare un assetto tra Stato e autonomie speciali improntato ad un maggior coordinamento sulle decisioni da assumere e sulle prerogative da rispettare. In particolare, nell'apposita indagine conoscitiva, deliberata il 25 febbraio 2015 e conclusa appunto con l'approvazione del documento finale nella seduta del 4 novembre 2015, si sono evidenziate criticità nel funzionamento delle Commissioni paritetiche, chiamate ad elaborare gli schemi di decreti legislativi di attuazione delle norme statutarie. Come detto, ciò rappresenta un terreno su cui promuovere una iniziativa al fine di realizzare una nuova stagione nei rapporti tra Stato e le singole autonomie speciali. Infine, signor Presidente, sul delicato tema dei rapporti finanziari, con riferimento ancora all'autonomia finanziaria delle Regioni speciali, la Commissione evidenzia l'opportunità di valorizzare l'esperienza di coordinamento infraregionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il sistema regionale integrato di finanza pubblica delineato in quella Regione può essere inteso per le autonomie differenziate come uno strumento di ricomposizione dei rapporti tra gli enti, a fronte della sostanziale mancata attuazione del disegno di federalismo fiscale previsto dalla riforma costituzionale del 2001 e sancito dal pluralismo autonomistico e dalla equiordinazione degli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli articoli 114 e 119 della Costituzione. Per quanto sopra esposto, il Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista esprimerà un voto favorevole sulla risoluzione proposta dalla relatrice.

abbiamo partecipato attivamente in tutte le sedute. Ringrazio la senatrice Orrù, che ha già ampiamente

l'ultima parte dell'intervento del sottosegretario Pizzetti, soprattutto perché egli rappresenta il Governo; due due giorni prima della festa della Repubblica, sentire un rappresentante del Governo che dice che la Repubblica non è solo lo Stato, ma è rappresentata dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali (Città metropolitane e Comuni) fa piacere, perché questo è un po' il cuore di questa indagine conoscitiva, cioè quello di ristabilire e cercare di armonizzare meglio i rapporti

Cogliendo una suggestione del senatore Quagliariello, quando parlava di un federalismo fiscale che è stato attuato a metà, faccio

effettivamente l'assetto del territorio e dello Stato si trova in difficoltà, perché tutta una serie di riforme legittime non si sono concluse.

Questa indagine, che la Commissione parlamentare ha voluto portare avanti proprio in seguito all'esito non confermativo del *referendum* costituzionale del 2016, ha inteso esaminare attentamente gli aspetti del rapporto tra lo Stato e gli enti della Repubblica, cercando di suggerire anche alcune soluzioni pratiche. Molti hanno enfatizzato la non attuazione dell'articolo 11 della riforma del 2001. Credo sia giusto

l'armonizzazione dei rappresentanti parlamentari in seno alla Commissione affari regionali con i rappresentanti delle Regioni, degli enti locali e dei Comuni.

non funzionano effettivamente così bene. C'è tutta una serie di criticità alle quali questa relazione cerca di dare delle soluzioni.

la Repubblica agli enti locali e alle Regioni, per dare maggiori possibilità ai territori.

del popolo italiano dello scorso 4 dicembre 2016 ha nuovamente posto all'attenzione dei costituzionalisti l'ormai decennale problema delle forme di raccordo fra Stato ed enti territoriali. Il superamento del bicameralismo perfetto e la configurazione del Senato quale Camera delle autonomie avrebbe consentito un più rapido ed efficace raggiungimento di posizioni condivise fra i diversi livelli territoriali, una semplificazione del quadro dei relativi rapporti ed il superamento del contenzioso istituzionale che ha subito un'implementazione notevole nel periodo postriforma del 2001. Credo che non si possa non convenire con i risultati a cui è giunta la Commissione bicamerale per le questioni regionali, che ha svolto un ottimo lavoro: l'unica soluzione percorribile per garantire una maggiore partecipazione degli enti territoriali al procedimento legislativo e, di conseguenza, avere benefici notevoli in tema di deflazione del contenzioso costituzionale, è quello di attuare la soluzione ponte che fu individuata nell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ossia l'attuazione di una Commissione bicamerale per le questioni regionali in forma integrata, che avrebbe consentito alla stessa di essere una sorta di laboratorio per il confronto istituzionale tra lo Stato e gli enti territoriali. È necessaria questa soluzione prospettata, perché il principio della leale collaborazione non deve costituire unicamente il cardine dell'attività degli esecutivi, ma anche il riferimento costante del legislatore. Le Assemblee parlamentari costituiscono, invece, la sede naturale per la realizzazione del principio di leale collaborazione, in quanto consentono di riportare nel circuito della democrazia rappresentativa l'adozione di scelte di fondamentale

interventi disorganici e disomogenei che spesso sono stati adottati senza l'inclusione nella discussione dei destinatari delle norme. Altro beneficio indiretto sarebbe la prevenzione del conflitto costituzionale tra Stato e Regioni. Il riparto di competenze legislative delineato dall'articolo 117 della Costituzione ha infatti ben presto dimostrato la sua insufficienza nella composizione degli interessi nazionali, regionali e locali. Con l'integrazione della Commissione bicamerale si consentirebbe di assicurare a monte del processo, nell'ambito del procedimento legislativo, il rispetto del quadro delle competenze L'integrazione della Commissione bicamerale, in ogni caso, non è sufficiente. È necessario delineare con precisione chirurgica anche i relativi competenze e poteri, soprattutto per evitare dannose sovrapposizioni con il sistema delle Conferenze, le quali costituiscono peraltro un luogo di concertazione degli esecutivi e non risultano la sede più appropriata laddove si tratta di incidere sulla funzione legislativa. Auspichiamo come Gruppo una rapida e proficua discussione di tutti i Gruppi in tal senso. Pertanto, voteremo a favore della relazione proposta dalla Commissione bicamerale.

il che non consente di "fare spallucce" di fronte a un'idea di riordino di tutta la materia, non solo sul piano dell'assetto democratico, ma sul piano proprio dell'equilibrio rispetto agli enti locali. È del tutto evidente, infatti, che la non presenza di voto direttivo e quindi di eletti a suffragio universale e la concomitante

al Presidente, che è il sindaco del capoluogo) ha determinato - lo dico in base a una breve verifica fatta in questi anni - indipendentemente dal colore politico, che l'*hinterland* di una grande città o addirittura di una metropoli è diventato il tappeto sotto cui mettere tutta la spazzatura. E quando parlo di spazzatura, molto spesso mi riferisco proprio alla spazzatura, perché è del tutto evidente che in assenza di un confronto democratico ogni problema di una città media, tanto più di una metropoli, troverà nella Provincia, nel territorio degli altri Comuni il luogo di risoluzione, non pagando prezzi di natura elettorale se non nello specifico Comune. Allora, qui doveva essere dato un segnale più forte. Ovviamente ci sono aspetti positivi che non ci sfuggono, come Sinistra Italiana, ma doveva essere dato un segnale più forte e, cioè, il pasticcio della legge doveva essere il primo aspetto ad essere affrontato in termini di cambiamenti profondi e di controtendenza legislativa profonda, perché altrimenti il rischio sarà che nelle prossime aperture di anno scolastico piuttosto che sul piano della viabilità e della difesa del territorio, che erano le competenze storiche delle Province tradizionali *ante*

come già ampiamente espresso nella discussione, le nostre perplessità sulla vaghezza di questo documento ci indurranno a esprimere un voto di astensione. Voglio solo aggiungere due motivazioni a questo voto di astensione, che vuole essere un incoraggiamento a trovare delle soluzioni per un migliore rapporto tra Stato e Regioni, ma anche una critica. Noi voteremo su un documento che impegna il Governo, per quanto di propria competenza, a dare corso alle indicazioni contenute nella relazione. Le indicazioni sono vaghe, quindi praticamente si sta dando al Governo la facoltà di scegliere tra le indicazioni scritte, alcune anche in contrasto,

che la superata specialità regionale voglia significare che non si è riusciti ad attuare appieno le forme di specialità regionale, tant'è che, come dice la relazione, addirittura ci sono Regioni come il Veneto e Lombardia che premono per andare verso una maggiore autonomia. Spero che su questo punto non ci sia un tornare indietro alle pretese di un *referendum* costituzionale bocciato, che tagliava tantissime competenze alle Regioni, perché per il polso che ho nelle Regioni a Statuto speciale,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione al nostro esame è il frutto del lavoro di una delle quattro indagini conoscitive svolte nell'ambito della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il lavoro della Commissione è iniziato e fortunatamente si è concluso con la stessa Carta costituzionale in quanto il *referendum* costituzionale del 4 dicembre è stato sonoramente bocciato e oggi non si può fare finta che le norme che prevedevano un enorme passo indietro sulle disposizioni disposizioni che riguardano le competenze delle Regioni non siano state respinte dagli italiani. Quindi, per fortuna, ci troviamo con la Costituzione vigente così come è stata modificata nel 2001, almeno nella parte che riguarda le autonomie regionali. iniziali a nostro avviso completamente sbagliate, innanzitutto perché nella riforma costituzionale proposta non c'erano le soluzioni ai problemi che hanno portato al contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni degli ultimi anni. Quindi, la risoluzione dei problemi passa anche dalla Commissione che ha redatto questa relazione. Tuttavia, per continuare a essere autorevole, dato l'alto compito che le è attribuito, tale Commissione non può prendere posizioni troppo sbilanciate politicamente, ma deve essere un organismo che lavora nell'interesse del titolo che le è proprio, proprio, appunto, per la risoluzione delle questioni regionali. Semmai, se proprio dobbiamo rimproverarci qualcosa come membri del Parlamento, lo dobbiamo fare rammaricandoci di non aver integrato prima, secondo le previsioni dell'articolo 11

tra i diversi livelli di governo. Sinora un luogo di compensazione delle controversie è certamente stato il complesso sistema delle Conferenze, fornendo un ruolo di supplenza rispetto alla mancata attuazione delle disposizioni di cui al citato

Abbiamo evidenziato che non siamo d'accordo sulle premesse, mentre possiamo esserlo sulle modalità di individuazione delle più opportune forme per integrare la Commissione per le questioni regionali con i rappresentanti delle autonomie. Così come si può trovare un percorso condiviso per il riordino del sistema delle Conferenze. Per quanto riguarda la revisione degli Statuti speciali, molte delle conclusioni della Commissione sono condivisibili, in quanto rappresentano un percorso di buon senso, che ovviamente deve essere condiviso con le stesse autonomie speciali. Nella prossima legislatura, chiunque vinca le elezioni, bisognerà anche fare tesoro di alcune indicazioni che emergono in questa relazione sul come integrare la Commissione per le questioni regionali. Così com'è sarà necessario studiare i modi per dare agli enti del territorio quell'autonomia di risorse che è il fondamento per inquadrarli nel modo più efficace nell'ambito di un regionalismo efficiente da tutti auspicato. concludere. Considerato che non condividiamo larga parte degli assunti di tipo politico della relazione, ma apprezziamo buona parte del lavoro istruttorio fatto in un consesso autorevole

per il lavoro che abbiamo fatto insieme e che lei in particolare ha curato presentandolo all'Assemblea, mi limiterò a svolgere due considerazioni. Quanto alla prima, è evidente che in esame, così come l'indagine conoscitiva ad essa sottesa avevano il compito di fornire al legislatore (quindi, in qualche modo, a noi stessi) alcune indicazioni di carattere regolamentare e, per alcuni aspetti, di carattere legislativo, al fine di intervenire a valle della mancata conferma della riforma costituzionale per dar corso a quanto contenuto nelle previsioni di cui all'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, rimaste lungamente in sospeso, anche nelle ultime legislature, in attesa della riforma, che peraltro la stessa legge costituzionale n. 3 indicava quale approdo conclusivo del processo riformatore delle relazioni e dei rapporti tra lo Stato e il sistema delle Regioni e delle autonomie locali. Da questo punto di vista, credo che sia l'indagine conoscitiva,

che anche le incompletezze e forse le mancanze di precisione nell'indicare alcuni punti debbano essere ricondotte al fatto che questa non era una relazione di accompagnamento a un disegno di legge - che non compete alla Commissione bicamerale per le questioni regionali

Sono molto d'accordo, peraltro, con la sollecitazione che veniva dall'intervento del sottosegretario Pizzetti, rispetto al fatto che, nella gamma delle ipotesi risolutive che la relazione propone, abbia un particolare rilievo il tema di come ricostruire un nesso, che poi è molto rilevante anche per il buon funzionamento delle istituzioni della democrazia, tra le funzioni e le competenze dello Stato e le funzioni e le competenze delle Regioni e degli enti locali. - di cominciare, soprattutto nell'integrazione della composizione della Commissione bicamerale, con l'assunzione, magari in una prima fase di carattere sperimentale, di quella rappresentanza delle Regioni e delle autonomie locali che era prevista nell'articolo 11 della legge n. 3 del 2001. Credo che questo sia il compito al quale, al di là dei diversi punti di vista che oggi si sono messi in gioco anche nella nostra discussione, dovremmo auspicabilmente cercare di lavorare per senso di responsabilità nei confronti del Paese e del funzionamento delle istituzioni democratiche, anche di quelle territoriali, che erano la *ratio* sottesa al tentativo di riforma costituzionale. è stato fatto un buon lavoro, che mette a disposizione di tutti noi strumenti su cui discutere (e mi auguro che si possa utilizzare anche la parte finale della legislatura per avviare questo tipo di lavoro),

si era affidato a un generoso tentativo di risolvere la questione trasformando questa Assemblea parlamentare in un'assemblea che avesse proprio il compito di assumere al massimo livello costituzionale le funzioni delle autonomie locali e delle Regioni in una sede parlamentare.

buttato alle ortiche - certamente con il responso inappellabile della maggioranza dei cittadini italiani - un'occasione che avrebbe potuto dare al regionalismo una sede istituzionale propria in cui esprimersi rappresenta un'occasione mancata, su cui dovremmo riflettere tutti quanti per cercare di superare positivamente, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, questo *gap*.